(Brusìo).* Colleghi, non si riesce nemmeno a parlare. Vorrei almeno essere messo in condizione di poter leggere: così non riesco a capire nemmeno quello che leggo. Comunico che in data 21 settembre 2009 è stato presentato il seguente disegno di legge: *dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell'interno*: «Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 2009, n. 131, recante ulteriore rinvio delle consultazioni elettorali amministrative nella provincia di L'Aquila»

Nel corso di questa settimana saranno discussi il decreto-legge recante disposizioni correttive del decreto anticrisi, il disegno di legge, già avviato, sull'istituzione di campi ormeggi attrezzati, nonché il disegno di legge sull'etichettatura dei prodotti agroalimentari e le ratifiche di accordi internazionali definite dalla Commissione. La prossima settimana, nella seduta pomeridiana di martedì 29 settembre saranno poste all'ordine del giorno le mozioni sul Fondo aree sottoutilizzate. Seguirà, a partire dal giorno successivo, l'esame del disegno di legge istitutivo del Ministero della salute ed eventualmente dei disegni di legge non conclusi.

A conclusione del dibattito il Presidente renderà le proprie comunicazioni ai sensi dell'articolo 126, commi 3 e 4, del Regolamento sul contenuto del disegno di legge finanziaria. Nel corso della stessa settimana si passerà poi all'esame del decreto-legge sul rinvio delle elezioni amministrative nella Provincia di L'Aquila. Nella settimana successiva, dal 12 al 16 ottobre, l'Assemblea non terrà seduta in relazione all'esame dei documenti finanziari da parte delle Commissioni. Infine, la Conferenza dei Capigruppo ha preso atto della proposta della Presidenza tendente ad introdurre una disposizione transitoria nel Regolamento al fine di dare soluzione alla questione posta dal Gruppo dell'Italia dei Valori circa la mancata presenza di un proprio rappresentante nel Consiglio di Presidenza. Una volta formalizzata tale proposta - auspicabilmente sottoscritta da tutti i Gruppi - la Presidenza si riserva di convocare la Giunta per il Regolamento fin dalla prossima settimana.

del decreto-legge n. 78 del 2009 recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali.

aggiunge il concerto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nelle decisioni del Consiglio dei Ministri in materia di interventi urgenti relativi alla trasmissione e alla distribuzione dell'energia, nonché di interventi riguardanti la produzione dell'energia. L'ulteriore modifica al comma 3 specifica che l'emanazione degli atti e provvedimenti, nonché di tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie all'autorizzazione e alla realizzazione degli interventi urgenti relativi alla trasmissione e alla distribuzione dell'energia, nonché di interventi riguardanti la produzione dell'energia sia effettuata dal Commissario quando le amministrazioni pubbliche non rispettino i termini previsti dalla legge o quelli più brevi fissati dallo stesso Commissario. Infine, con una modifica al comma 4-*quater*, viene eliminata la previsione della nomina dell'amministratore delegato della società Stretto di Messina spa a commissario straordinario delegato, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge n. 185 del 2008, sostituendola con la previsione della nomina di un commissario straordinario senza ulteriori specificazioni. La seconda modifica concerne l'articolo 13-*bis*. L'integrazione apportata al comma 3 chiarisce che dall'ambito applicativo delle disposizioni in materia di scudo fiscale rimangono esclusi i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto legge. Infine, all'articolo 17 si modifica il comma 30-*ter*, dove si ribadisce che l'esercizio dell'azione di danno erariale da parte delle procure della Corte dei conti è esercitabile a fronte di una specifica e concreta notizia di danno. Inoltre, si chiarisce che il corso della prescrizione dell'eventuale illecito contabile rimane sospeso fino alla conclusione del procedimento penale. Un'ulteriore modifica apportata al comma 30-*quater* ribadisce l'esclusione della colpa grave quando il fatto dannoso tragga origine dall'emanazione di un atto vistato e registrato in sede di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti precisa che tale esclusione rileva solo relativamente ai profili dell'atto già esaminati in sede di visto di legittimità. Anche in questo caso, non vi sono osservazioni di carattere finanziario da formulare alla luce dell'eliminazione dalla norma di possibili limiti all'esercizio dell'azione di danno erariale. modifiche che ho brevemente sintetizzato non sono da considerare uno stravolgimento del decreto approvato lo scorso luglio, quanto piuttosto opportune razionalizzazioni. Opportune perché finalizzate ad integrare la portata di alcune norme di quel testo, completandone e precisandone aspetti tecnici, ma anche - e forse principalmente

sollevando polemiche ovviamente comprensibili da un punto di vista politico, ma a mio avviso un tantino ridondanti. Si tratta di un'opportunità che il Governo ha ritenuto tale anche in seguito alle considerazioni svolte dal Presidente della Repubblica, in sede di approvazione del decreto-legge n. 78 del 2009, circa le disposizioni sulla Corte dei conti. Il dibattito sviluppatosi nel corso dell'esame in sede referente - che ritengo sostanzialmente, anzi, profondamente proficuo, soprattutto per l'apporto di alcuni esponenti della Commissione bilancio (come il senatore Morando, il senatore Lusi anche il senatore Lannutti) - ha mantenuto questa impostazione, riuscendo a far emergere e ad evidenziare i contenuti effettivi del provvedimento, chiarendo quei rilievi considerati criticità e ritagliando inoltre qualche profilo di ulteriore precisazione. A questo proposito, vorrei evidenziare che le modifiche di cui stiamo parlando, in fondo, sono di fonte parlamentare: si sono rese possibili perché il Parlamento ha svolto il proprio ruolo, quindi derivano dalla discussione e dal confronto - anche serrato - di opinioni diverse, quale hanno avuto modo di realizzare le Commissioni 5a e 6ª riunite in occasione del loro esame. Le sempre richiamate prerogative del Parlamento si sono pertanto sviluppate in un dibattito utile e costruttivo. Al di là dei giudizi critici espressi dall'opposizione su "come" il Governo abbia deciso di correggere il precedente decreto-legge n.

Per inciso, ritengo che quel "come" non corrisponda ad una confusione legislativa, come qualcuno l'ha voluta definire, ma ad un normale apprezzamento di opportunità da parte dell'Esecutivo nel formulare e sottoporre al Parlamento provvedimenti che attengono alla propria responsabilità. Con riferimento allo scudo fiscale, la discussione ha consentito di dire chiaramente che non si tratta di riciclaggio di Stato, come pure è stato definito dal senatore Lannutti con parole tanto comprensibili quanto foriere di sovrabbondanti polemiche. Lo scudo, infatti, non è un'iniziativa estemporanea del nostro Governo con annesso un effetto di spiazzamento in favore di chiunque, furbetti residenti in paradisi fiscali o meno: è un'iniziativa, vorrei ricordarlo, che deriva da una strategia definita a livello internazionale proprio per combattere questa tipologia di paradisi - e magari indirettamente evitare ulteriori scossoni al sistema finanziario internazionale - nel contesto dell'impegno volto a promuovere una più ampia riforma del sistema stesso. Non è molto lontana la richiesta del presidente Obama all'UBS (Unione delle banche svizzere) di allentare il segreto bancario per far rientrare denari americani nel proprio Paese; non è nemmeno lontano l'accordo Gran Bretagna-Lussemburgo per l'operazione definita «*New disclosure opportunity»*, che tra l'altro qualche giornale ha scoperto solo ieri - vedi il "Corriere della Sera"

il messaggio che questo Governo lancia a quegli evasori, ai furbetti, a chi ha voluto portare all'estero risorse che, se investite in questo Paese, ci avrebbero aiutato ed oggi ci aiuteranno - noi confidiamo - nell'affrontare la crisi Sembrano peraltro essere state fugate le riserve espresse in merito ad altri aspetti evidenziati come critici. Le recenti disposizioni attuative emanate in queste settimane dall'Agenzia delle entrate (anche se ancora in bozza ed oggetto di consultazione) ribadiscono l'interpretazione fornita nel corso della discussione e sulla quale il Governo aveva concordato come, ad esempio, l'attuazione mediante il rinvio alla versione precedente dello scudo, l'anonimato, la copertura per le violazioni tributarie e previdenziali, l'impraticabilità del rimpatrio e della regolarizzazione nelle more di accertamenti in corso. disposizioni, nonostante l'apparente complessità, fanno dello scudo uno strumento importante che, come scriveva qualche tempo fa un grande economista, già Ministro delle finanze, Francesco Forte, risponde alle classiche massime fiscali: il tributo deve essere semplice, certo e fornire un buon gettito. È esattamente questo che il nostro Governo si attende. Vorrei altresì evidenziare come lo scudo costituisca un'occasione per riflettere su alcuni decisivi argomenti, peraltro correlati; l'occasione per riflettere sulle motivazioni economiche che, non da sole, spingono a portare fuori i capitali; l'occasione per rivedere il rapporto fisco-contribuente sulla base di regole e comportamenti più trasparenti ed equi per ciascuna delle parti; l'occasione per ribadire la necessità di un'efficace lotta all'evasione e all'elusione, specialmente nei periodi di difficoltà, per far rientrare quelle risorse che, insieme ad altre, consentano consentano di perseguire l'obiettivo strategico di ridurre il carico tributario e la pressione fiscale, obiettivo che è sempre presente nei nostri programmi e nella nostra azione di governo. A tal proposito, mi sembrano importanti non solo i dati forniti dal direttore dell'Agenzia delle entrate in un convegno di qualche giorno fa, ma anche l'idea dello scudo come cerniera nella lotta all'evasione, nonché le sue dichiarazioni sulla complessiva attività di accertamento, che stanno a dimostrare la convinzione con la quale il Governo intende portare avanti questa sfida. L'occasione, insomma, per riflettere sulle indicazioni lasciateci da un importante studioso come Ezio Vanoni, anch'egli Ministro delle finanze, che negli anni Cinquanta credeva in un rapporto di reciproca fiducia fra contribuente e fisco, e nel fatto che la riduzione delle imposte dovesse essere accompagnata da uno scambio di natura etica: minori tasse in cambio di maggiore sincerità nel pagamento delle imposte. Mi sembra, invece, ci siano adeguati margini per una precisazione sul ruolo dei professionisti nelle procedure di rimpatrio e regolarizzazione alla luce delle vigenti norme antiriciclaggio: una lacuna di queste prime disposizioni attuative - peraltro non sanabile autonomamente dall'Agenzia delle entrate - che potrebbe essere colmata proprio in questa sede parlamentare, poiché questo Parlamento ne è stato investito dai territori**,** dai rappresentanti delle categorie e, soprattutto, degli albi professionali Per quanto riguarda le disposizioni relative alla Corte dei conti, ricordo che sono proprio le polemiche seguite all'emanazione delle disposizioni di cui all'articolo 17, commi 30 e seguenti, del decreto-legge che hanno in parte contribuito a intraprendere la strada della correzione o, meglio, della precisazione sui contenuti di quelle norme e sul fatto che non vengono in alcun modo depotenziati ruolo e funzioni della Corte dei conti. Anche in questo caso la discussione in Commissione ha contribuito a risolvere i dubbi interpretativi ed a giungere a conclusioni sulle quali il Governo si è dichiarato d'accordo. A proposito delle condizioni per l'azione di danno erariale della magistratura contabile, è stato evidenziato come essa fosse condizionata dall'esistenza di una notizia di danno definita troppo genericamente «specifica e precisa» e

l'unico significato possibile delle norme è quello di evitare che vengano aperti procedimenti che non abbiano poi un reale fondamento, ma che tanto danno fanno alle nostre amministrazioni in generale e, in particolare, a quelle che più ci stanno a cuore, vale a dire alle amministrazioni locali e al loro funzionamento.

valgono cioè per i prossimi procedimenti. Peraltro, non è stato sufficientemente evidenziato come la nullità prevista dalle norme vigenti non valga *ope legis*, ma sia lasciata ai possibili interessati e come venga conservata alla Corte la decisione di accettare o meno la sollevata eccezione di nullità. Vorrei ricordare, inoltre, che il decreto pone in capo alla Corte dei conti il potere di perseguire anche il danno all'immagine della pubblica amministrazione, elevando così a rango normativo una figura finora solo giurisprudenziale, la cui applicazione è analoga di cui all'articolo 17, sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

si possa leggere anche in senso estensivo. In altre parole, ritengo che ci possano essere i margini per interventi chiarificatori non solo "nelle" norme contenute nel proprio la sede di un provvedimento di necessità ed urgenza consente di prevedere norme che estendono la portata di quelle originarie e di esplicitarne il contenuto. È il caso, ad esempio, dei richiamati obblighi dei professionisti nelle procedure dello scudo. Allo stesso modo, si potrebbe presentare la necessità di estendere il contenuto anche di altre parti del decreto-legge, per precisarne e renderne più chiare portata e finalità, ed è quanto auspico in questa discussione generale. il relatore Gentile di competenza della Commissione finanze e tesoro del Senato, è composto da due soli articoli, di cui uno relativo all'entrata in vigore. presenta una serie limitata di interventi correttivi al decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, nel testo convertito dalle Camere, il cosiddetto decreto anticrisi. Dette modifiche scaturiscono, secondo quanto si evince dalla premessa del provvedimento, dalla ritenuta straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure correttive del suddetto decreto. La relazione illustrativa del disegno di legge di conversione chiarisce che l'intervento con decretazione d'urgenza è finalizzato a superare in radice possibili dubbi interpretativi o evitare i rischi derivanti, in sede applicativa, da formulazioni talvolta equivoche quanto al rispetto delle attribuzioni istituzionali delle diverse amministrazioni coinvolte. Poiché l'intento del Governo è quello di evitare l'entrata in vigore delle norme oggetto di modifica nel testo approvato con la legge di conversione, il decreto-legge in esame è entrato in vigore il giorno 5 agosto 2009, contemporaneamente alla legge di conversione del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, che va a modificare. Le modifiche apportate dal decreto riguardano i seguenti ambiti: innanzitutto la concertazione fra tutti i Ministri interessati, nonché i poteri del Commissario nominato dal Consiglio dei ministri in materia di interventi urgenti relativi alla trasmissione, alla distribuzione e alla produzione di energia; in secondo luogo, la nomina del Commissario straordinario delegato della società Stretto di Messina spa; luogo, i poteri di intervento della Corte dei conti in materia di danno erariale; infine, lo scudo fiscale introdotto dall'articolo 13-*bis* del decreto-legge n. 78 del 2009. Per quanto riguarda, in particolare, questo ultimo intervento, la lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 1 del provvedimento in esame modifica il comma 3 dell'articolo del decreto legge n. 78 del 2009, con il quale è stata introdotta nel nostro ordinamento una disciplina in materia di emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero mediante la procedura del rimpatrio ovvero della regolarizzazione (il cosiddetto scudo fiscale). Il citato comma 3, in particolare, ha disposto che il rimpatrio o la regolarizzazione non possono costituire elementi utilizzabili a sfavore del contribuente in ogni sede amministrativa o giudiziaria, in via autonoma o addizionale. Con la modifica apportata dal testo in esame se ne chiarisce in senso restrittivo la portata applicativa, precisando che sono escluse dall'applicazione delle suddette disposizioni i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto-legge. Rispetto a questo provvedimento, le Commissioni 5a e 6a riunite in queste settimane (dall'8 settembre in poi) hanno lavorato alacremente per apportare ulteriori modifiche.

In sintesi, una prima modifica è intervenuta al citato comma 3 dell'articolo 13-*bis*, precisando che il rimpatrio o la regolarizzazione non possono costituire elemento utilizzabile a sfavore del contribuente, in ogni sede amministrativa o giudiziaria, civile, amministrativa ovvero tributaria, in via autonoma o addizionale. Una seconda modifica è intervenuta anch'essa al comma 3 al fine di limitare gli obblighi di segnalazione previsti all'articolo 41 del decreto legislativo n. 231 del 2007, normativa di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio. Una terza modifica ha riguardato il secondo periodo del comma 4 e, per effetto di essa e per l'applicabilità degli articoli 14, 15 e 17 del decreto-legge n. 350 del 2001, con il pagamento dell'imposta diventa applicabile quanto previsto dall'articolo 1, comma 6,

diretto ad estendere alle imprese estere, controllate o collegate, l'applicabilità della disciplina dello scudo fiscale. In tale ipotesi, gli effetti del rimpatrio o della regolarizzazione si producono in capo ai partecipanti limitatamente agli importi delle attività cui è stato applicato lo scudo

nell'Aula dal Senato e siamo disponibili ad ogni contributo, così come avvenuto in Commissione, su alcuni emendamenti. Ritengo poi di poter ringraziare il Governo, rappresentato dal sottosegretario Giorgetti e la collega Bonfrisco per il lavoro svolto in queste settimane. *(Applausi

il decreto-legge al nostro esame nasce dalla straordinaria necessità ed urgenza di impedire che entrassero in vigore alcune delle norme del decreto legge anticrisi di luglio. il relatore è stato di una onestà cristallina nel fare questa affermazione, perché le norme che la maggioranza e il Governo hanno tentato di introdurre con questo decreto-legge sono oggettivamente delle correzioni del decreto-legge anticrisi di luglio. Non v'è chi non veda, dai resoconti parlamentari delle Commissioni 5a e 6a e dell'Aula, che queste che queste cose erano già state abbondantemente dette dai banchi dell'opposizione, con dovizia di particolari, su questi tre temi e su altri. È dovuto intervenire il Quirinale - la nostra massima Quirinale - la nostra massima carica istituzionale, il Presidente della Repubblica - ad imporre all'Esecutivo l'approvazione di un decreto-legge due giorni prima della promulgazione della legge di conversione del decreto anticrisi affinché modificasse queste tre norme. E anche su questo, signor Presidente, la maggioranza

Allora, chiunque abbia l'onore e il privilegio di essere seduto su questi scranni ha il dovere di contribuire a migliorare le norme che sono parte dell'ordinamento vigente. Voi avete iniziato questo processo di miglioramento con la proposizione di questo decreto-legge. Ciò nonostante siete riusciti nella fase di conversione qui, nel Senato della Repubblica, ad ulteriormente emendare tale provvedimento con norme che francamente sono in parte decisamente peggiorative del testo iniziale.

in merito al contenuto dell'articolo 13-*bis,* novellato da questo decreto-legge, e l'ulteriore modifica che solo oggi pomeriggio le Commissioni riunite hanno avuto modo di leggere, licenziata grazie al voto della maggioranza, sulla annosa questione della utilizzabilità dello scudo fiscale relativamente ai procedimenti in corso? Vede, signor Presidente, il fatto che si stia ragionando all'interno della maggioranza su come riuscire a districarsi in materia di applicabilità di questo provvedimento ai procedimenti in corso è cosa ormai nota: la settimana scorsa ci proponete di renderlo applicabile anche ai procedimenti penali; questa settimana ci dite, invece, che è applicabile soltanto a quelli civili, amministrativi e tributari, salvo inserire però,

abrogata con una legge del 2005? Perché, in realtà, l'operazione di quel procedimento del 2002 non è definitivamente conclusa. Allora voi pensate di introdurre con questa norma un ulteriore intervento nella sede penale che certo non migliora.

all'esclusione - una volta introdotto lo scudo - dell'obbligo di denuncia da parte dei professionisti per le normative antiriciclaggio:

di applicare in modo positivo e non in termini giuridici le maggiori entrate derivanti da questo provvedimento, e allora avete ristretto i termini per l'utilizzabilità di questo scudo, facendone terminare l'applicazione al 15 dicembre 2009. Avete cioè compreso che fare cassa poteva essere utile invece che rinviare, come sempre, all'ultimo momento; non si capisce però perché alcuni passaggi della

avendo come fonte legislativa il solo articolo 13-*bis* in oggetto. Mi riferisco, signora Presidente, onorevole Sottosegretario, signori relatori, alla numerosa casistica inserita in questa circolare, resa pubblica

sto facendo l'avvocato di nessuno, sto soltanto dicendo che quando a luglio vi abbiamo detto che c'erano numerosi problemi, e li abbiamo elencati uno per uno, non avete avuto il coraggio e l'umiltà di accettare i nostri consigli. Oggi ci proponete all'approvazione

che permettono ai nostri uffici finanziari di conoscere quanto i cittadini italiani fanno in determinati Stati esteri oltre l'Unione europea e lo spazio economico europeo. Mi riferisco al decreto del ministro Amato del 4

che svolgono attività finanziarie di carattere societario o patrimoniali in Stati diversi da quelli dell'Unione europea e dello spazio economico europeo. Sto parlando delle *white* *lists*, signora Presidente,

finale sarà che quei patrimoni, quei fondi, quei capitali, quelle attività finanziarie realizzate con società all'estero attraverso fondi transitati per via non legittima resteranno lì, non emergeranno. Le casse dello Stato non ne avranno beneficio perché nessuna imposta sarà

luglio 2009, n. 78, convertito con legge 3 agosto 2009, n. 102, fu modificato una prima volta dal Governo con un maxiemendamento, per recepire gran parte delle integrazioni introdotte dai colleghi deputati. Successivamente, con il decreto-legge che oggi siamo chiamati ad approvare, il Governo ha ritenuto necessario apportare altri aggiustamenti al decreto-legge n. 78, giustificati dalla straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure correttive per superare possibili dubbi interpretativi. Quindi, le correzioni sono state apportate soprattutto per chiarire e per meglio specificare, come i relatori hanno già affermato. Poiché l'intento del Governo era quello di evitare che entrassero in vigore norme di dubbia interpretazione, comunque approvate nel testo del decreto-legge n.

Questo è il senso politico di una scelta che ha destato inutili polemiche estive e comiche accuse di attentato alla democrazia da parte del Governo. Abbiamo trascorso l'estate balneare a parlarne.

Il decreto, infatti, non contiene alcun intervento sulla cosiddetta tassa sull'oro (intervento che è stato sollecitato da varie parti, anche a livello europeo), in quanto - come ha precisato in una nota il Presidente del Consiglio - è stato ritenuto sufficientemente chiaro il testo contenuto nella legge n. 102. Di fatto, a proposito della Corte dei conti, il nuovo disegno di legge prevede che «le procure della Corte dei conti possono iniziare l'attività istruttoria ai fini dell'esercizio dell'azione di danno erariale a fronte di specifica e concreta notizia di danno, fatte salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge». Inoltre, per quanto concerne il danno di immagine, nella relazione illustrativa è stato chiarito che «il corso della prescrizione dell'eventuale illecito contabile resta sospeso fino alla conclusione del procedimento Si risponde così a chi paventava la paralisi dell'azione della magistratura contabile, che certamente nessuno vuole e nessuno ha pensato di realizzare. Al Ministero dell'ambiente è stato riconosciuto di avere un ruolo, di concerto con gli altri Dicasteri interessati, nelle procedure per realizzare le grandi opere energetiche e infrastrutturali, comprese le nuove centrali. All'articolo 13-*bis*, comma 3, del decreto-legge n. 103 del 2009 viene chiarito, a proposito dell'operazione per il rientro dei capitali introdotta alla Camera, che i procedimenti in corso per fuoriuscita dei capitali all'estero non saranno fermati dallo scudo fiscale previsto dal decreto anticrisi. Nessun favore

procedimenti aperti con la giustizia, a riprova che questo Governo persegue solo gli interessi generali del Paese e non concede favori a qualcuno. Il decreto‑legge in esame oggi elimina poi il riferimento all'amministratore delegato della società Stretto di Messina spa La modifica, come ribadisce anche la relazione governativa, va a sottolineare il carattere generale della previsione normativa, al fine di evitare il possibile equivoco interpretativo legato alla circostanza secondo la quale un intervento volto ad assicurare l'avvio delle attività connesse alla realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina potesse essere invece ricondotto esclusivamente alla nomina, in qualità di commissario delegato, Ritengo dunque che questa opera del Governo, volta a recuperare chiarezza interpretativa ad un decreto abbondantemente modificato per recepire quanto stabilito dalla Camera dei deputati, sia certamente sostenibile e non alcun *vulnus* alle procedure costituzionali, vista anche la contestualità, richiesta dalla Presidenza della Repubblica e opportunamente attuata dal Governo,

come dimostrano anche i segnali di ripresa che già vengono rilevati dagli indicatori economici e, soprattutto, dalla fiducia delle famiglie, dei cittadini e del popolo italiano.

L'eccezione alla regola, però, ci viene offerta da questo Governo. In fondo, se questo provvedimento fosse stato corretto approvando gli emendamenti che noi avevamo presentato durante la sua conversione in legge nel mese di luglio,

Sostanzialmente il Governo, con lo scudo fiscale, ha fatto rientrare dalla finestra ciò che aveva allontanato dalla porta principale.

maggioranza introduce una correzione alla correzione, prevedendo l'impossibilità di utilizzare le prove ricavate dal rientro dei capitali dall'estero nei procedimenti penali in corso, e allarga l'esclusione della punibilità Credo che questo sia un fatto che deve farci riflettere molto (poi passerò ad affrontare brevemente un altro argomento). Credo che dopo

proprio sul tema del comportamento dei parlamentari molto si sta dicendo e molto ci si sta spendendo in questi mesi e in questa legislatura. Purtroppo voi accettate l'illegalità come regola

la maggioranza dei quotidiani ha riportato i dati del fallimento che sta facendo registrare il decreto di regolarizzazione delle colf e delle badanti.

Sostanzialmente voi avete fatto in modo che oggi in Italia continui a sussistere e a persistere l'irregolarità.

*(IdV)*. Signora Presidente, signor Sottosegretario, signori relatori, onorevoli colleghi, il decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103, recante disposizioni correttive

solleva delle questioni con il Presidente della Repubblica, poiché nel mese di agosto il presidente Napolitano fece cambiare la norma per evitare un'amnistia su procedimenti in corso.

pone, per noi dell'Italia dei Valori che abbiamo a cuore la legalità e la difesa dei diritti, problemi molto importanti.

«Con l'amnistia fiscale, 100 miliardi di euro stanno per tornare in Italia e le banche italiane e svizzere sgomitano per acchiapparne una fetta. L'Italia,» - spiega il quotidiano americano - «alla ricerca di denaro per colmare il deficit, lancia un'enorme amnistia sui capitali portati all'estero per sfuggire alle tasse». Anche Gran Bretagna e Germania hanno di recente lanciato amnistie ma, osserva il quotidiano finanziario, quella dell'Italia è la terza in sette anni - e mi scuserà l'ottima relatrice, senatrice Bonfrisco, se io continuo a definirla un riciclaggio di Stato - e sarà di gran lunga la più grande. In palio ci sono ben 100 miliardi di euro, stando alle attese del Governo, e gli evasori fiscali che si mettono in regola devono pagare una penalità di appena il 5 per cento di quello che vogliono dichiarare. E le loro identità restano segrete. È l'amnistia più favorevole ai contribuenti di quanto contemplato in qualsiasi altro Paese. Nelle precedenti amnistie le banche svizzere sono state le vincitrici. *Credit Suisse* è riuscita a mantenere dal 60 all'80 per cento dichiarati dagli italiani spostandone gran parte in nuove filiali in Italia. UBS, l'Unione banche svizzere, ne ha mantenuti il 50 circa 6 miliardi di euro, alimentando la spinta a diventare la più grande banca estera privata in Italia. Ma ora le banche svizzere sono sulla difensiva a causa dell'erosione del segreto bancario le banche italiane sono decise a competere. In passato offrivano pochi prodotti d'investimento, oggi invece stanno migliorando le loro offerte, si stanno mobilitando, lavorando in stretto contatto con quei fiscalisti che sono stati citati citati dai relatori, organizzando seminari per i clienti e istruendo i loro esperti sugli intrighi dell'amnistia fiscale. Si offrono di prestare agli investitori le somme da pagare per le multe scontando le loro commissioni.

riunite - né desta meraviglia che primarie banche italiane ed internazionali truffino il fisco italiano. Ciò che è stupefacente è che il Ministro dell'economia e delle finanze continui ad affidare a queste banche, accusate di frode fiscale, le operazioni di collocamento titoli e *bond* italiani sui mercati internazionali invece di depennarle dalla lista degli istituti di credito di riferimento del Tesoro. Forse perché vi sono complicità e legami che non possono essere recisi. Ora, su questa amnistia, su questo scudo allargato, intervengono tante operazioni. Voglio ricordare l'operazione in gergo denominata "*easy risale al 2005, quando, dopo un'indagine sulle richieste di rimborso inoltrate da società inglesi, il nucleo repressione frodi della Guardia di finanza di Roma trasmise un rapporto alla procura di Pescara, competente per territorio, riportate grandi banche internazionali, come Lehman Brothers, Goldman Sachs, JP Morgan, Banca Intesa, Deutsche Bank, Citybank, che avevano frodato il fisco italiano per un controvalore di 4,3 miliardi di euro. Il 5 maggio puntualmente, tramite il lavaggio dei dividendi, veniva chiesto il rimborso.

una grande *performance*. Le società Goldman Sachs e Jp Morgan sono state attivissime. E così via. Sul banco degli imputati di quell'operazione ci sono le case madri e le filiali europee di queste grandi banche. sono pesantissime: dalla truffa ai danni dello Stato, tentata e consumata, alla responsabilità penale e amministrativa per non aver adottato misure idonee tendenti ad evitare

champagne. Comprendo che ci sono commercialisti come, tra quelli che sono stati ricordati, Tommaso Di Tanno, uno dei maggiori tributaristi italiani e già presidente del collegio sindacale di diverse grandi aziende, tra cui BNL, Vodafone, Omnitel e attualmente in quello di Monte dei Paschi di Siena, che che sono a favore di questo scudo allargato. Voglio però ricordare che ci sono anche altre operazioni in atto da parte delle procure della Repubblica e della Guardia di finanza. Mi riferisco all'operazione Brontos. Senatrice Bonfrisco, lei che ha una competenza molto approfondita in merito a quello che sto dicendo, comprende quello che sto affermando.

A Londra è scoppiato il finimondo, ma da noi non accade nulla: in pochi hanno notato che uno dei sette *dossier* riservati coinvolgeva due banche italiane: Unicredit e Intesa. Si chiama progetto Brontos ed è tutto molto semplice: i banchieri brinderanno questa sera o domani con lo champagne. Mi avvio alla conclusione, signora Presidente, visto che il tempo sta terminando. La pacatezza e la competenza del sottosegretario Giorgetti così come le dotte relazioni dei relatori, la senatrice Bonfrisco e il collega Gentile, non ci fanno cambiare opinione in merito ad una sanatoria, un condono tombale che rappresenta uno schiaffo alla moltitudine dei contribuenti onesti, quella moltitudine che manda avanti la baracca e fa il proprio dovere con il fisco. Si tratta di un paracadute per i troppi furbetti del quartierino, per quei banchieri che ho ricordato, per quei riciclatori di denaro sporco che hanno di che brindare. Noi non siamo d'accordo e voi ci permetterete

euro per regolarizzare un collaboratore domestico ed infine le procedure *on line* particolarmente complesse. Questi tre aspetti nell'ordine del giorno da noi presentato si accompagnano ad un'altra proposta, che per noi rappresenta il nodo politico che fin dall'inizio abbiamo

la possibilità di adottare un apposito provvedimento volto ad estendere la possibilità di aderire alle dichiarazioni di emersione del lavoro irregolare a chiunque occupi alle proprie dipendenze cittadini privi di titolo di soggiorno

«Le difficoltà legate alla crisi avvertite dagli italiani possono aver determinato anche un calo del livello di tolleranza nei confronti degli immigrati, come dimostra l'aumento degli episodi di discriminazione, il 22,1 per cento dei quali subiti in ambito lavorativo: il 32,1 per cento delle denunce riguarda la fase di accesso al mercato del lavoro, il 23,2 per cento le condizioni lavorative, il 19,6

Sono stati fatti provvedimenti importanti per contenerlo e ridurlo e far sì che ci sia più trasparenza nei confronti della società civile da parte del mondo del credito. Voglio anche ricordare, a questo riguardo, l'intervento che ha voluto il ministro Maroni nel costituire osservatori regionali

vorrei invece riprendere alcuni di questi temi che hanno più interesse e vicinanza con il mondo delle autonomie locali, al quale mi sento particolarmente legato, come amministratore e sindaco di una città,

che riguardano il sistema tributario e contabile, che sono di esclusiva competenza delle Regioni (questo provvedimento è assolutamente rispettoso per quanto riguarda questo profilo) e anche la materia dell'energia, che invece è di competenza concorrente. apprezziamo e riteniamo importante quanto previsto in questo provvedimento, che restituisce anche centralità e attenzione agli enti locali, Grazie,

alla sezione centrale il controllo di legittimità su molti atti, specialmente di assegnazione di consulenze e quant'altro. Alcune spese che riguardano la loro potestà autonoma devono rimanere nell'ambito del controllo esercitato a livello locale. Capiamo che questo possa eventualmente

a chiarire e ad estendere il ruolo centrale delle autonomie locali e regionali. L'auspicio è che sia sempre più tenuto in considerazione il livello regionale, per quanto riguarda l'energia, estendendo tale ruolo anche agli enti locali,

Signora Presidente, signor Sottosegretario, quando quest'estate si è discusso, col decreto-legge anticrisi (il n. 78 del 2009), dell'introduzione dello scudo fiscale, intervenendo in Aula avevamo avuto modo di stigmatizzare il provvedimento, forti della convinzione che, se si vuole davvero condurre una battaglia ferma contro l'evasione fiscale, il primo principio da affermare è quello di non acconsentire ad alcuna ragione per giustificare l'operato di chi ha preso e prende in giro la legge. a maggior ragione dopo che già ad inizio decennio, fra il 2002 e il 2004, si era fatto ricorso per due volte a scudi. Lo Stato deve perseguire chi evade, non premiarlo: invece si continua a mortificare i tanti, tantissimi contribuenti leali, lavoratori dipendenti, pensionati, professionisti autonomi, piccole e medie imprese, mentre si strizza l'occhio complice a chi si è prodotto in gravi e sanzionabili violazioni delle norme tributarie. C'è il fondato sospetto che in tutto questo tempo di gran parlare dello scudo che sarebbe arrivato, e con criteri sempre più tolleranti e permissivi, si sia di fatto ulteriormente incentivata la fuga di capitali all'estero. Della serie: siccome si sa che la sanatoria ci sarà, e si può presumere che le norme saranno al solito lasche, portiamo in fretta fuori quello che poi si potrà regolarizzare a prezzi di saldo, come puntualmente sta avvenendo. In questo quadro, sinceramente avvilente, era venuto almeno il parziale conforto della misura disposta con il decreto-legge correttivo del 3 agosto 2009, n. 103, anche in ossequio a provvidi suggerimenti venuti dalla Presidenza della Repubblica: si escludevano dalla possibilità di accesso allo scudo le situazioni interessate da provvedimenti sanzionatori in corso alla data del 5 agosto 2009, così da non vanificare il tanto lavoro degli uffici delle Entrate e della Guardia di finanza, oltre che di altri attori istituzionali, impegnati seriamente e con brillanti risultati nel contrasto all'evasione su scala internazionale e verso i cosiddetti paradisi fiscali. Ma oggi, con le modifiche introdotte dagli ultimi emendamenti, la situazione si aggrava in modo clamoroso. L'estensione della non punibilità penale per molti profili di reati societari e contabili per effetto dello scudo, rende sempre più simile il provvedimento a un vero e proprio condono generalizzato; e questa ulteriore e pesantissima forzatura disvela - se ancora ce n'era bisogno tutta la mistificazione delle pretese di collocare lo scudo fiscale in salsa italiana nell'ambito di quella vasta azione intrapresa da diversi Stati nei confronti dei paradisi fiscali. Questo è ciò che il ministro Tremonti, il Governo e la vostra maggioranza - lo ha sottolineato anche nel suo intervento la relatrice, senatrice Bonfrisco - ci vorrebbero far apparire. Ma la realtà, a ben vedere, è molto, molto diversa. Perché, anziché costituire un atto di battaglia contro l'evasione fiscale e i paradisi fiscali e condurre una lotta a muso duro, fianco a fianco, insieme ai principali *partner* europei e americani, se si analizzano comparativamente le procedure, le somme da versare e le regole sull'anonimato, si vede che il nostro, o meglio il vostro scudo fiscale sembra fatto apposta per favorire i contribuenti infedeli; con buona pace dell'ineffabile Ministro dell'economia che, nelle interviste che rilascia in Italia e in Europa, continua impudentemente ad affermare che lo scudo fiscale britannico, per esempio, sarebbe di gran lunga più conveniente e permissivo di quello italiano. Niente di meno vero: se si guarda cosa prevedono, punto per punto, gli scudi fiscali varati da Stati Uniti, Francia e Gran Bretagna, la differenza è abissale ed è tutta a vostro disdoro!

ricordato che, se fossero stati regolarmente dichiarati, per quei 100 euro di redditi evasi si sarebbero dovute pagare imposte ordinarie intorno ai 43 euro. In aggiunta, va sottolineato che il ritardo con il quale l'Italia procede nella rinegoziazione degli accordi con i paradisi fiscali intenzionati ad uscire dalla *black list* dell'OCSE ne compromette il risultato. Per uscire da quella lista, i Paesi in essa presenti devono rinegoziare accordi di scambio di informazioni con almeno 12 Paesi. In molti casi le negoziazioni si sono concluse o sono in corso con un numero di Paesi superiore a 12. dunque da temere che, quando sarà il turno dell'Italia, il nostro potere negoziale risulterà infimo, dato che l'obiettivo del Paese-paradiso fiscale sarà già stato raggiunto. Ed è proprio tale atteggiamento rinunciatario che dà ragione del costo così modesto chiesto per la sanatoria all'evasore italiano, perché tanto più efficace è la negoziazione ed ampio il varco che si apre nel segreto bancario, tanto più forte è l'effetto deterrenza, per cui si può pretendere un onere maggiore da chi chiede la regolarizzazione. Invece, ancor più per effetto dell'estensione dei salvacondotti che si è voluto ulteriormente introdurre, il provvedimento che discutiamo si connota, anche al di là dell'entità del gettito che potrà derivarne, col profilo di un sostanziale condono ad amplissimo spettro. Ed è altrettanto chiaro che, così facendo (lo dico con amarezza), si produce un ribaltamento nel sistema dei valori, rendendo la tutela dei «colletti bianchi» privilegiata rispetto ai principi di civiltà, di equità e di trattamento paritario verso tutti; con quale danno per i già malmessi e bistrattati spirito civico, senso di responsabilità e interesse generale di questo Paese lascio a voi immaginare. Così, oltre al danno, si aggiunge la beffa. Prima sono stati cancellati i principali provvedimenti antievasione (conti correnti dedicati per le attività economiche e professionali, divieto di pagamento in contanti, assegni non trasferibili: tutto svanito). Poi sono state ridotte le sanzioni. Adesso c'è un condono a prezzi di saldo. E così la giostra dell'evasione riprende a girare sempre più veloce. Lo confermano purtroppo anche i dati del calo delle entrate nei primi sette mesi del 2009, che cresce rispetto al 2008, e in cui continua una flessione del gettito dell'IVA (del 6 per cento, quasi 6 miliardi di euro, ormai già oltre il livello del dato finale 2008), che non pare essere correlabile con il modificarsi della tipologia dei consumi delle famiglie, certo più orientate a prodotti essenziali ad IVA più bassa, ma probabilmente compensato dalla crescita del numero delle famiglie. Insomma, signor Sottosegretario, insisto a sottolinearlo: permane e si consolida quella sfasatura tra il forte calo dell'IVA e la decelerazione assai più contenuta dei consumi, che è spia, molto concretamente, proprio della tendenza a crescere dell'evasione. Da ultimo, poiché via via anche le scuse nobili di condonare gli evasori al fine di far ritornare i capitali condonati in Italia e sostenere gli investimenti delle imprese in una difficilissima fase di crisi o di destinare le risorse di gettito alla ricostruzione dell'Abruzzo trovano scarse condizioni di garanzia e praticabilità, ed emerge sempre più l'imperativo di far cassa senza guardare troppo per il sottile, a conferma che i conti tanto in ordine poi non sono, mi permetto di avanzare in conclusione qualche modesta proposta, forse utile a riscattare almeno in parte la negatività del provvedimento. Penso a come potrebbe essere sensato destinare quota parte del gettito ricavato, se significativo, a ridurre, se non strutturalmente, almeno *una tantum* la pressione fiscale su redditi da lavoro e pensioni, magari anche solo intervenendo sulla detassazione delle tredicesime, soprattutto per le fasce di reddito più basse, come vi avevamo invano sollecitato a fare come Partito Democratico già l'anno scorso. E se proprio lo stato della finanza pubblica è così in sofferenza (ma ci dovreste spiegare dove sono andati a finire quei 35 miliardi dì maggiori spese nell'anno corrente), almeno fate il bel gesto di finanziare, per l'anno 2010, la messa a regime del 5 per mille, premiando con un riferimento certo quel volontariato che svolge una funzione indispensabile di sussidiarietà, di sussidiarietà, non solo per la solidarietà verso i deboli, ma anche in termini di coesione sociale. So che non se ne farà niente, ma invito il ministro Tremonti a pensarci seriamente: dopo essere passato in un solo anno da sedicente Robin Hood a un più prosaico venditore, senza principi e ideali, di indulgenze a potenti ed evasori, corroborare lo spirito del 5 per mille con un po' di risorse potrebbe almeno servirgli, se non da esimente, a schivare qualche pesante ironia e insofferenza la prossima volta che ci intratterrà con dissertazioni sull'etica e i massimi principi della responsabilità e del rigore nella gestione dell'economia e della finanza. *(Applausi

In particolare, tutto questo si inserisce in uno scenario che vede ancora il nostro Paese ad un livello di tassazione pari

anche il fardello dei due anni successivi allo scudo fiscale precedente, quello di un Governo che di colpo ha aumentato la tassazione dal 41 al 43 per cento e che ha creato la fuga dei capitali dal nostro Paese. Ci troviamo nella condizione di avere un debito pubblico di molto superiore al PIL e anche quel 43 per cento di tassazione è in realtà ben più alto, perché tutti noi ci rendiamo conto del livello di evasione nel quale anche in ambito nazionale ci veniamo a trovare. coloro che pagano le tasse pagano ben più del 43 per cento di media; la media tra i soggetti pagatori probabilmente va oltre il 50 Con una situazione che ben ha tradotto il ministro dell'economia, Tremonti, in cui i dati del bilancio dello Stato e il debito pubblico ampiamente superiore al PIL non ci permettono di fare *deficit* perché perderemmo di credibilità e i costi economici e di conseguenza sociali sarebbero tali da non essere sopportabili per il nostro Paese. Da qui le azioni che è possibile fare in questo momento di grande transizione, verso - come tutti speriamo - una ripresa economica generale, senza perdere di vista anche il disegno generale

che devono determinare un nuovo modello di Stato (vorrei ricordare la legge sul federalismo fiscale e quindi la sua attuazione nei prossimi anni, la legge di riforma della contabilità dello Stato) e quindi un sistema che inciderà fortemente sulla gestione delle risorse pubbliche. È proprio in questo momento che dobbiamo svolgere tali azioni perché

i creditori che sono molti cittadini italiani. Il debito pubblico probabilmente verrà pagato con il rapporto rispetto al prodotto interno lordo (e allora, dovremo farlo salire)

sul cosiddetto scudo fiscale con la sua duplice azione. Non c'è dubbio che una prima azione sia quella di portare fondi alle casse dello Stato, senza aumentare la tassazione ai cittadini italiani e prendendo da coloro che non hanno subito, probabilmente, tassazione in passato. Ma la seconda azione, che io reputo più importante, di natura macroeconomica, è quella di portare nel Paese capitali che vengano spesi ed investiti.

forzato sulle depenalizzazioni, lo dico francamente. Se un'azione deve essere fatta, deve essere chiara e trasparente. L'emendamento del collega Fleres in Commissione ha fatto fare un passo avanti già notevole. Mi auguro che il Governo, nei suoi indirizzi anche all'Agenzia delle entrate e agli organi di controllo, permetta di emanare un sistema di norme amministrative e di attuazione che creino il massimo di chiarezza: quella chiarezza che in questo momento (me ne sono reso conto anche dal dibattito in Commissione) non c'è in modo completo.

L'azione del Governo e del Parlamento, la nostra azione, il nostro dovere è di creare le condizioni per attrarre capitali nel Paese perché, se portiamo il Paese ad essere in grado di attrarre capitali,

Governi di centrodestra e di centrosinistra dobbiamo avere il coraggio di leggere la realtà economica, sociale e dei tempi e anche delle tecnologie che stiamo vivendo. Oggigiorno, se guardiamo ai dati delle dichiarazioni e alle produzioni dei redditi, con le moderne tecnologie e la mobilità delle persone che la realtà moderna e gli strumenti moderni permettono, i redditi sono trasferibili ovunque con estrema facilità e in tempo reale.

Che senso ha ancora la progressività delle imposte dirette quando poi, nel confronto con la realtà, notiamo che questa colpisce solo alcuni? Colpisce cioè tutti coloro che per l'entità dell'importo,

ma anche della riforma delle imposte dirette, per introdurre un modello di tassazione che probabilmente non può che essere legato ai consumi; se infatti siamo in un mercato comune vedo quanto mai difficile andare a rincorrere il singolo: si tratta di andare a rincorrere l'oggetto. Questo penso debba essere l'oggetto investire ancora questa legislatura; deve essere un modello che andrà a fare il paio con la riforma federalista del Paese.

ripresa, a intervenire sull'emergenza di quei vagoni che con la ripresa probabilmente non ripartiranno con la locomotiva: il treno ripartirà, ma non tutti i vagoni ripartiranno. ripartiranno. Sappiamo che il Governo è pronto, che gli stessi fondi dello scudo sono destinati in gran parte agli interventi di carattere sociale,

ai colleghi intervenuti nell'ambito di questa discussione, sia durante l'esame delle Commissioni 5a e 6a riunite, così come in quello ancor più interessante avvenuto in quest'Aula, vorrei poter replicare con molta chiarezza

il ruolo meritorio che l'opposizione ha avuto nell'affrontare la discussione di questo decreto correttivo. Così come nessuno di noi si è dimenticato che questo decreto correggeva

del Presidente della Repubblica e - io dico - anche da altre parti, quando si era appunto fatto notare, durante la discussione avvenuta prevalentemente alla Camera,

della grande e profonda crisi finanziaria che ha originato questa crisi economica, che ormai pervade l'economia reale non solo del nostro Paese, che è anche uno dei pilastri fondamentali su cui si giocherà la possibile ripresa, la possibile uscita da questa crisi, cioè quello del credito e delle banche, voglio ricordare voglio ricordare che, sia nella Commissione finanze del Senato, sia - anche più ampiamente - in altri settori delle nostre istituzioni, della politica e del Governo, il tema delle banche è considerato sensibile e importante. Non potrebbe che essere così, del resto, e non solo in relazione all'etica dei comportamenti, così come sono emersi da quel poco o quel tanto che conosciamo degli aspetti più

la nostra e la mia attenzione, perché so che non è lì la soluzione dei problemi. Occorre invece trovare il modo di evitare, scongiurare in futuro le orribili e devastanti speculazioni che hanno visto le banche protagoniste di una stagione economica particolarmente infelice,

del confronto tra politica, istituzioni e banche certamente è e sarà dura, difficile e che quei colletti bianchi non devono essere guardati con alcuna forma di riguardo da parte di nessuno di noi (e non mi pare che il Governo faccia questo), ma che forse è difficile per la politica essere forte e con la schiena diritta davanti alle soluzioni proposte dai banchieri,

l'ambiguità non serve in questo momento. Mi riferisco soprattutto a quei senatori che parlavano di confusione del Governo negli interventi legislativi. di un normale apprezzamento di opportunità da parte del Governo nel formulare e riproporre al legislativo provvedimenti che attengono alla propria responsabilità. Così come eviterei, caro collega Lannutti, di parlare di riciclaggio di Stato con riferimento alle norme sullo scudo fiscale. Capisco bene la polemica e la dialettica politica, ma non facciamoci del male da soli con

con effetto di spiazzamento in favore dei furbetti residenti nei paradisi fiscali, ma è una scelta che deriva da una strategia internazionale, volta proprio a combattere i paradisi fiscali

attraverso le dichiarazioni riservate agli intermediari, che garantiscono l'anonimato delle dichiarazioni di emersione delle attività nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Vorrei inoltre fare una l'anonimato favorirebbe in qualche modo la criminalità organizzata. Credo che questa sia una *boutade*, o forse vi è un pizzico di ingenuità da parte del senatore Lannutti. L'intermediario finanziario conosce bene persone ed aziende e quindi, a mio giudizio, commetterebbe consapevolmente un reato se operasse il rimpatrio o la regolarizzazione di disponibilità derivanti da attività criminose o illegali. Un'ultima considerazione sullo scudo. scudo. Io mi pongo una domanda, e credo se la pongano tutti gli uomini di buon senso: se dovesse fallire il rientro di questi danari, dovremmo tutti interrogarci sui motivi per i quali lo Stato non riesce ad attrarre e a far ritornare le proprie risorse. questo il vero tema sullo scudo fiscale, che non interessa - come sapete - i poveri cristi, ma interessa larghi patrimoni portati all'estero da persone che hanno grandi disponibilità finanziarie.

Cari colleghi, cari amici, non c'è stata la norma *extralarge* e non c'è stata nemmeno la norma *large*: si è ritornati allo scudo del 2002. Mi auguro che questo scudo abbia la possibilità di far rientrare

debbano essere agevolate in qualche modo, perché ad oggi mi sembra uno scudo abbastanza incagliato (per usare un termine bancario). Facciamo dunque in modo (tutti assieme i legislatori di questo Stato) che

volute dall'opposizione e dal Governo e, quindi, pienamente condivise, con pieno riconoscimento da parte dell'opposizione di quella che era stata una richiesta accolta.

luogo quello di garantire un percorso di rientro di capitali dall'estero a vantaggio del tessuto produttivo nazionale e di un sistema che complessivamente abbiamo cercato di attivare attraverso una serie di provvedimenti

È evidente che quando il Governo ha deciso di adottare lo strumento dello scudo fiscale ha fatto una scelta politica molto precisa, quella di attivare comunque tale strumento

ben conoscendo i temi affrontati ma, soprattutto, la chiusura, che noi riteniamo essere già significativa a livello politico, svolta in Commissione.

Esaminati altresì gli emendamenti ad esso riferiti esprime, per quanto dì competenza, i seguenti pareri: - parere non ostativo sull'emendamento 1.203, segnalando l'opportunità di un coinvolgimento delle Regioni in relazione alla definizione delle modalità per la formazione e la certificazione professionale degli addetti in materia di trasporto fluviale,

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo ad eccezione delle proposte 1.3, 1.2, 1.38, 1.49, 1.200, 1.203, 1.208, 1.62, 1.204 e 1.205, sulle quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione».

nelle sedi opportune, iniziative utili a rappresentare alla BCE l'opportunità di istituire un gruppo di lavoro finalizzato al contrasto del riciclaggio del denaro e dell'evasione fiscale». Così riformulato, l'ordine

la data per la regolarizzazione delle badanti al 31 ottobre. Ciò consentirebbe

prevedendo il non pagamento per la badante e, invece, il pagamento per la colf. La scelta discende dalla constatazione che chi assume la cosiddetta badante non lo fa per scelta, ma per necessità;

Al tempo stesso, con l'emendamento 1.200 per le colf o collaboratrici domestiche prevediamo la possibilità di cumulare le ore presso diversi datori di lavoro, cosa che oggi non è possibile. Questi punti sono stati evidenziati dalle associazioni sindacali, dalle associazioni dei datori di lavoro ed anche dalle associazioni che si occupano del fenomeno migratorio e quindi riscontrano l'unanimità

mi permetto di richiamare l'attenzione del Governo su questo tema e mi auguro che in un successivo provvedimento sia possibile trovare anche la copertura necessaria a integrare quella disposizione che in sé è giusta, ma che rischia di penalizzare una parte importante di lavoratori e di piccole e medie imprese.

va ribadita la nostra contrarietà all'intero complesso dell'iniziativa relativa allo scudo fiscale, e particolarmente all'integrazione e all'ampliamento

l'articolo 3 del decreto-legge n. 78, alcuni commi del quale prevedono di poter utilizzare i certificati verdi (che sono uno strumento di incentivazione espressamente finalizzato a promuovere le fonti energetiche rinnovabili) per l'energia prodotta attraverso sistemi di cogenerazione non necessariamente legati all'uso di rinnovabili. Quindi, di fatto, essi configurano un utilizzo abusivo ed improprio dei certificati verdi, in qualche modo

uno contro l'altro utilizzi energetici entrambi virtuosi, ma che devono poter contare su meccanismi di incentivazione certi, credo sia una scelta errata, che già un precedente Governo Berlusconi aveva fatto e sulla quale peraltro era dovuto ritornare perché si era reso conto di aver penalizzato il mercato delle rinnovabili; mercato che, negli ultimi mesi, in Italia ha conosciuto, malgrado

uno dei più discussi e discutibili. Si tratta dell'articolo che prevede la possibilità di decidere che per determinate opere pubbliche, infrastrutture energetiche in particolare, si ricorra a procedure decisionali e autorizzative abbreviate attraverso la nomina di un commissario. Non c'è dubbio che questo decreto correttivo

a mia firma, di cui uno soppressivo dell'articolo 4 e gli altri correttivi, chiedono comunque di intervenire su una norma che rimane ancora molto discutibile e criticabile. Ciò innanzitutto perché lascia a tre o quattro Ministri la scelta di decidere quali opere e quali infrastrutture energetiche debbano poter accedere alle procedure commissariali in maniera del tutto discrezionale, visto che in essa non sono sostanzialmente definiti i criteri per tale Inoltre, il concerto delle Regioni è previsto per le infrastrutture di produzione dell'energia, ma non per quelle di trasmissione e distribuzione della stessa.

numerosi contenziosi tra lo Stato e le Regioni. Ne consegue che anziché accelerare le procedure per la realizzazione di opere di trasmissione e distribuzione di energia, essa rischia di rallentarle ulteriormente. Resta molto vaga la necessità per il commissario di attenersi alle procedure fissate in sede europea per ciò che riguarda la VAS, la VIA, l'IPPC. Inoltre,

o di tipo storico, artistico e monumentale) possano essere aggirate o comunque se ne possa tener conto in misura meno cogente di quanto preveda la normativa, in questo caso, nazionale. I tre emendamenti 1.10, 1.18 e 1.24, in maniera più o meno generale, tendono a porre rimedio

Il problema centrale che questi emendamenti, sia pure con modulazioni e graduazioni diverse, vogliono porre all'attenzione dell'Aula e dei rappresentanti del Governo è quello di una compartecipazione, di una corresponsabilizzazione e di una condivisione delle scelte nel settore importante e vitale dell'energia da parte degli enti locali e dei Comuni.

compartecipazione degli enti locali alle decisioni sull'energia. Ciò non riguarda quindi soltanto l'individuazione dei siti di produzione,

avevamo assistito a diverse formulazioni di semplificazione delle scelte in campo di politica energetica del nostro Paese. scelte, presentate come la necessità di una semplificazione e di un decisionismo, in realtà avevano determinato una *deregulation*, una totale deregolamentazione della necessità di porre la tutela dall'ambiente e della salute pubblica come punto prioritario di una qualsiasi politica del Governo nazionale.

di quel fenomeno che proprio questa mattina Tito Boeri, in un interessante articolo, ha definito «il federalismo alla rovescia», un federalismo di annunci e di proclami, in cui di fatto i Comuni, che dovevano essere i protagonisti del federalismo delle autonomie, sono sistematicamente messi da parte. Lo abbiamo visto con l'abolizione dell'ICI, dell'ICI, con il blocco dell'IRPEF e dell'IRAP, e lo abbiamo visto con la ripartizione dei fondi FAS. Oggi si perpetua ancora una volta una totale totale messa da parte delle responsabilità degli enti locali e dei Comuni nelle decisioni che riguardano la politica energetica. Né possiamo credere, come è stato replicato in Commissione bilancio, che queste scelte

come ha ricordato il senatore Della Seta, e non si capisce quali siano gli obiettivi e le finalità che il Governo si propone. l'assenza di un piano energetico e una totale disattenzione nei confronti degli Accordi di Kyoto per quanto riguarda il potenziamento delle energie rinnovabili.

modulati e graduati a seconda della necessità di raggiungere un tentativo di intesa con la sensibilità di alcuni componenti della maggioranza,

legittimità. Alla luce dell'abolizione di qualunque forma di controllo preventivo sugli atti degli enti locali, in applicazione della legge costituzionale n. 3 del 2001,

8.000 Comuni, nel momento stesso in cui devono affidare un incarico anche di piccola entità, debbono mandare gli atti alla sezione centrale della Corte dei conti: sono stati eliminati i controlli regionali per poi attuarne uno a livello centrale.

All'articolo 2, comma 2, viene introdotto un meccanismo corretto. Per accelerare il superamento della commissione di massimo scoperto, questo provvedimento introduce una norma che pone a carico delle imprese lo 0,5 per cento di spese generali:

una dichiarazione se non addirittura una garanzia di impunità ed un invito a delinquere in materia fiscale e tributaria. Stiamo parlando dell'estensione dello scudo fiscale

Tali modifiche sono finalizzate ad ampliare in maniera del tutto impropria i meccanismi di tutela a favore dei soggetti che effettuano operazioni di rimpatrio o regolarizzazione delle attività finanziarie detenute all'estero. Basta ricordare le

Ma c'è anche il punto 2) che, per certi versi, è ancora più grave perché stabilisce che il pagamento dell'imposta comporta l'esclusione della punibilità, ovviamente da un punto di vista penale, per tutta una serie di reati. Innanzitutto, per reati in materia tributaria, poi per reati contro la fede pubblica e privata e per reati in materia societaria. Mi limito ad elencare alcuni di questi reati, per renderci conto compiutamente di cosa si va a modificare. I reati per i quali viene esclusa la punibilità sono la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fattura e altri documenti, la dichiarazione fraudolenta mediante artifici, dichiarazione infedele, omessa dichiarazione, occultamento o distruzione di documenti contabili. Gli altri reati contro la fede pubblica o privata sono i reati di falso indicati in questa esclusione di punibilità. Infine, ricordo i reati in materia societaria che sarebbero esclusi dalla punibilità e che sono quelli relativi alle false comunicazioni sociali e alle false comunicazioni sociali in danno delle società, dei soci e dei creditori. L'ultimo punto, il 4), amplia gli effetti della sanatoria non soltanto ai soggetti privati

gli effetti del rimpatrio si producono anche in capo ai partecipanti, nei limiti degli importi delle attività rimpatriate, e quindi, anche in questi casi, si esclude la punibilità sotto il profilo penale per reati commessi fino al 31 dicembre 2008. In questo senso, riteniamo molto grave la previsione di questa garanzia di impunità e di questo invito a delinquere. Il secondo emendamento che voglio presentare è l'1.40, che fa riferimento alla materia concernente la procura generale e l'attività delle procure presso la Corte dei conti. Si tratta dell'articolo 17 del decreto-legge anticrisi, che modifica il comma 30*-ter* e il comma 30*-quater*. Innanzitutto ricordo (e ne riparleremo anche in sede di dichiarazione di voto) che vi sono evidenti profili di illegittimità costituzionale, da noi già segnalati nella discussione che abbiamo svolto precedentemente. Ora vengono proposti alcuni correttivi, peraltro molto limitati, prendendo atto di alcune considerazioni formulate anche all'interno della Commissione giustizia di questo Senato e, in misura e in maniera molto garbata, anche dal Servizio studi del Senato. Voglio ricordarvi di cosa si tratta, perché qui si interviene sulla possibilità, per il magistrato della procura contabile, di agire in assenza di una notizia di danno, che deve essere però qualificata in maniera molto particolare in quanto si parla di notizia specifica e concreta. A nostro parere, come segnalato già all'interno della Commissione

che in questa materia aveva distinto, in maniera molto precisa e corretta, tra la necessaria previsione della richiesta di atti e documenti in sede di attività istruttoria da parte del procuratore contabile rispetto alla notizia di danno, che può essere anche formulata in maniera ipotetica a seconda delle segnalazioni che pervengono all'ufficio del procuratore contabile. Qui c'è confusione, non si sa se voluta o meno, rispetto a questi due concetti:

alla necessità di intervenire in sede di correzione del decreto-legge n. 78 su una norma o sulla interpretazione di questa norma che sta destando moltissima preoccupazione tra le persone portatrici di handicap.

a determinare il blocco delle assunzioni di personale presso le pubbliche amministrazioni, appare infatti una disposizione che sembra riferire questo divieto di autorizzazione ad assunzioni anche alle assunzioni di carattere speciale. Si ritiene - così hanno ritenuto molte amministrazioni pubbliche - che tra le assunzioni di carattere speciale siano ricomprese quelle previste dalla legge n. 68 del 1999, cioè le assunzioni delle persone portatrici di disabilità per le quali la legge dispone il collocamento obbligatorio. Nelle scorse settimane effettivamente diverse pubbliche amministrazioni, avendo così interpretato la norma, hanno bloccato processi di assunzione già programmati, con ciò destando grande sconcerto e preoccupazione nelle persone

riguardi anche le categorie speciali, cioè i soggetti portatori di disabilità. La situazione del collocamento obbligatorio di queste persone versa già in condizioni di particolare difficoltà perché la situazione di crisi economica in cui versano molte aziende sta ovviamente rallentando e sostanzialmente bloccando i percorsi di inserimento lavorativo dei soggetti disabili. Questo determina ovviamente, oltre che una limitazione dell'esercizio di un diritto alla piena integrazione lavorativa e sociale, anche il rischio di costi economici e sociali certamente molto pesanti per l'intera collettività. quindi al Governo la disponibilità a rivedere le disposizioni previste nel decreto n. 78 o comunque a chiarirne il dispositivo, precisando quali debbano essere in questa materia i comportamenti della pubblica amministrazione a tutela del diritto al lavoro dei disabili e delle persone con limitazione della autonomia.

per la valorizzazione dei ricercatori. Questa Aula e quella della Camera ha sentito ripetutamente parlare, anche da parte del Ministro competente per materia, della necessità di valorizzare i ricercatori, che quando si trovano in momento professionalmente molto proficuo proficuo rischiano di essere appunto rottamati. Chiediamo quindi di aggiungere a tale norma, oltre ai magistrati, ai primari ospedalieri ed ai professori universitari, anche i ricercatori universitari.

prima svuotare e poi rinviare l'azione di classe. Domani alle ore 10,30 ci sarà una manifestazione delle principali associazioni dei consumatori davanti a Montecitorio, cui aderisce la Coldiretti, anche per chiedere un ripensamento da parte del Governo su questa azione collettiva. Basta leggere i giornali: il Governo si lamenta dell'arroganza e della protervia delle banche.

Como 150.000 euro per la continuità aziendale. Oggi un altro imprenditore, Antonio Mangone, di 42 anni, ha messo un'inserzione

come sappiamo, prevede la possibilità per la pubbliche amministrazioni di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro a decorrere dal compimento dell'anzianità contributiva di quarant'anni. Poco tempo fa, come ha detto prima la senatrice Garavaglia, la legge n. 15 del 2009 aveva invece chiarito che il diritto di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro competesse alle autorità della pubblica amministrazione solo per i dipendenti con 40 anni di servizio effettivo. Ripeto, è una legge del 2009. A pochi mesi di distanza, si

con un'età magari inferiore ai 60 anni, in piena controtendenza, cari colleghi, rispetto all'andamento generale europeo e anche italiano dell'azione di pensionamento. Non dimentichiamo poi la delicatezza di un *top down*,di un atto dirigistico nei confronti di una data fondamentale per il *planning* di vita, come è la data di pensionamento. La data di prevedibile prevedibile pensionamento è fondamentale nella vita di una persona, non la si può sovvertire con un *top down* in questo modo. L'emendamento 1.74 propone

Esprimiamo un giudizio severamente critico nei confronti della misura dello scudo così come è stata concepita e per come si è via via sviluppata fino all'ultima formulazione. Ribadisco che consideriamo che lo Stato dovrebbe affermare il rispetto della legalità e non avere atteggiamenti in qualche modo permissivi nei confronti di chi le leggi le disattende e in qualche caso anche le irride.

entrate e la situazione economica generale può portare a considerare l'utilità di un provvedimento di carattere eccezionale, ma siamo alla patologia di tali provvedimenti. È il terzo scudo fiscale nell'arco di un decennio per cui quelli che già si erano avvantaggiati nelle due precedenti situazioni, se si ritrovano oggi in una condizione analoga,

dell'eticità e dello spirito pubblico. Sono valori di cui il Paese avrebbe bisogno per affrontare la crisi e per fare coesione sociale tanto quanto le risorse di carattere economico-finanziario per sostenere gli investimenti per lo sviluppo. Muoversi in questa direzione certamente determinerà, alla lunga, un danno complessivo per il gettito, per i comportamenti generali e non genererà al contrario tante risorse per compensare questi elementi di negatività.